L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico.

e colpito l'intera Nazione, ma che riguardano sempre la questione della manutenzione delle autostrade italiane. Parliamo di arresti da parte della magistratura dopo una lunga indagine. Questo ovviamente non può non interferire con l'interrogazione e anzi la rende ancora più attuale, alla luce degli ultimi avvenimenti che comunque sono inquietanti e sui quali abbiamo chiesto specifiche informazioni al Governo in questa Aula.

per riprendere il controllo del sistema autostradale italiano; un prezzo esorbitante anche per i ripetuti annunci fatti persino da esponenti del Governo, che hanno provocato nei mesi scorsi diversi fenomeni borsistici e che qualcheduno addirittura ha definito operazioni di aggiotaggio. In secondo luogo, l'azione dello stesso Governo, che poche ore fa, prima degli arresti, ha comunque esteso il *golden power*, cioè lo scudo che il Governo può porre di fronte a scalate ostili che vengono dall'estero, proprio sul settore autostradale; una coincidenza che denota ed evidenzia quanto importante sia la questione.

uno di essi è famoso nel mondo per le speculazioni che fa a danno degli utenti e a esclusiva remunerazione degli azionisti, esattamente come Atlantia.

pochi giorni fa, un tunnel in Virginia, guarda caso dal fondo australiano che dovrebbe acquistare le azioni in Italia, per un miliardo di euro. Chiedo quindi al Governo quali sono i tempi dell'operazione per consentire ai cittadini italiani di riprendere il possesso del sistema autostradale del Paese, affinché esso risponda davvero agli interessi nazionali degli utenti, e quali sono gli investimenti necessari per garantire l'assoluta manutenzione, per riparare a una ferita che non riguarda solo la città di Genova, ma l'Italia intera.

della relazione della commissione insediata dal precedente Governo, che aveva ritenuto la procedura di revoca sottoposta a numerose problematicità per motivi giuridici. Tale relazione - come sapete - è pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A seguito dell'insediamento dell'attuale Governo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia hanno proseguito negli approfondimenti sulle proposte che la società Aspi e successivamente anche Atlantia hanno fatto al Governo per superare, ed eventualmente transare, la richiesta di revoca. Il 14 luglio il Consiglio dei ministri ha esaminato queste proposte e ha avviato un *iter* formale di definizione della transazione, su presupposti sostanziali e non formali di interesse pubblico, che sono legati esattamente alla questione delle manutenzioni (sulle quali poi peraltro tornerò tornerò alla fine, senatore Urso), alla quantità e alla mole di investimenti necessari alla rete autostradale e alle attività connesse, nonché basati sull'esigenza di garantire i livelli occupazionali, soprattutto in un momento così così faticoso per il nostro Paese. A seguito di questo, ovviamente, si è aperto da una parte l'*iter* transattivo con il Ministero delle infrastrutture, la Presidenza del Consiglio e il MEF, per quel che riguarda la costruzione del piano economico-finanziario (il cosiddetto PEF), che dovrà avere l'approvazione finale di vari soggetti

una trattativa formale con Atlantia per l'acquisizione della maggioranza della società Aspi. Sul fronte della trattativa tra Cassa depositi e prestiti e Aspi, il mio Ministero non ha ma posso rappresentarle che tale trattativa si muove su prezzi e valori di mercato, in termini prospettici, e non incrocia altre decisioni che questo Governo dovrà prendere a breve. Per quel che riguarda, invece, la questione delle manutenzioni e la vicenda delle indagini di ieri, non voglio sottrarmi

gennaio 2020, controlli effettuati da terzi. Terzo: linee guida uguali per tutti, concessionari e gestori, sulla sicurezza di ponti e di viadotti stabilite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici a gennaio 2020. Quarto: quadruplicamento delle multe per tutti gli inadempimenti minori propri sul fronte delle manutenzioni. Tutto questo, senatore Urso, ha portato in questo anno a centinaia di milioni di euro di cantieri da parte di tutti i concessionari; per me, cantieri urgentissimi che hanno creato disagi e fiumi di polemiche. Alla luce dei fatti, confermo la bontà di quella scelta. non posso che giudicare la risposta, purtroppo, anche agli occhi degli italiani e non soltanto delle famiglie delle vittime o della città di Genova, inadeguata e direi anche evasiva sui tempi e sulle modalità che debbono consentire al nostro Paese di riprendere il controllo di ciò che, come è evidente a tutti anche dall'inchiesta giudiziaria in corso, è sfuggito ad ogni controllo. La città di Genova è stata ferita, ma non piegata. Sono passati oltre due anni. Lei stessa ha parlato del settembre del 2018: siamo ormai a novembre del 2020: sono passati oltre due anni. Il Governo non è cambiato. La guida del Governo è sempre del *premier* Conte, che ha cambiato parere diverse volte questo periodo di oltre due anni, e del MoVimento 5 Stelle, che è il partito di maggioranza relativa allora come oggi. oggi. Per questo noi ci riteniamo assolutamente insoddisfatti della risposta, che non chiarisce nulla, tantomeno sull'ipotesi che intervenga un fondo straniero che prenderebbe il controllo della società, e che nel suo comportamento è stato giudicato, dagli inglesi che l'hanno subito, come un fondo vampiro, un canguro vampiro che succhia il sangue degli utenti, il denaro e le risorse senza investire. Rischiamo di cadere dalla padella alla brace. Mi stupisco che, nella maggioranza chi per primo ha sollevato la questione oggi resti silente. Per questo, la nostra risposta, che è la risposta della Nazione italiana a un Governo inadempiente, è sicuramente: purtroppo avete perso oltre due anni e non ci dite quando chiuderà questo *affaire*. Perché di questo ormai si tratta, di una straordinaria operazione finanziaria

il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, il cosiddetto conto termico, la cui disciplina è stata aggiornata con decreto interministeriale del 16 febbraio 2016. Le modalità di accesso al conto termico, così come definite nel decreto interministeriale citato, sono molto stringenti e limitate al solo imprenditore agricolo professionale, escludendo di fatto numerose piccole aziende agricole, in particolare quelle maggiormente presenti nelle aree interne e montane. interne e montane. La qualifica di imprenditore agricolo professionale stretta a colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro per cento per le aziende ubicate in zone svantaggiate) e che per ottenere tale qualifica, rilasciata dall'amministrazione competente (Regione o Provincia autonoma), è necessario essere iscritti alla gestione agricola dell'INPS. Nei territori montani però molti agricoltori non possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale perché, a causa del basso reddito agricolo, sono costretti a lavorare anche fuori della loro azienda. Tuttavia per le aziende agricole dei territori delle aree interne e montane, anche di piccole dimensioni, l'interesse verso l'installazione di sistemi innovativi di riscaldamento a biomassa è molto elevato visto il risparmio di costi che ne deriva, ampliare la platea dei beneficiari degli incentivi previsti dal conto termico anche alle imprese agricole il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile sarebbe anche in perfetta sintonia con quella politica *green* tanto auspicata e sostenuta livello europeo e condivisa dal nostro Governo. Si chiede perciò se il Ministro in indirizzo condivida l'opportunità di tale ampliamento, che significa anche incrementare la percentuale di impiego di fonti energetiche rinnovabili, con ricadute positive sulla sostenibilità ambientale e, in caso affermativo, se non intenda intervenire direttamente in tal senso apportando le necessarie modifiche al testo del decreto interministeriale del 16 febbraio 2016.

l'accesso alle aziende agricole definite, come giustamente diceva il senatore interrogante, «imprenditore agricolo professionale». Ricordo che tale disposizione però deriva dal dettato normativo europeo secondo il quale possono godere delle sovvenzioni comunitarie le sole aziende agricole in grado di dimostrare redditività. Quindi il legislatore, e in questo caso il Ministero che ha fatto una norma di secondo livello, si è riferito all'articolo 2135 del codice civile proprio perché lì c'è la dimostrazione della redditività. Infatti, il decreto legislativo n. 99 del 2004 ha previsto che l'accesso fosse legato all'essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, al dedicare all'attività agricola almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e, soprattutto, al fatto che i ricavi da tale attività fossero almeno il 50 per cento del proprio reddito. nelle zone montane questa percentuale è ridotta al 25 per cento, dando quindi una più ampia possibilità agli agricoltori di essere considerati come imprenditori agricoli professionali. Condivido ovviamente la necessità di promuovere ogni forma di

discussione debba essere fatta anche sulla base di un'analisi costi-benefici perché il conto termico, di fatto, è costituito da soldi che vengono prelevati dalle bollette, quindi, a ogni aumento di disponibilità del conto termico e a ogni ampliamento della platea corrisponde una ricaduta sulla bolletta. Va fatta con grande attenzione un'analisi costi-benefici di tutte le possibilità di ampliamento di accesso al conto termico e certamente questo è uno dei temi che potrà essere valutato con maggiore attenzione.

in futuro si possano prendere anche delle misure concrete per l'agricoltura interna e di montagna, che è una delle filiere più importanti

*(IV-PSI)*. Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sappiamo tutti che il 31 ottobre scorso lo stabilimento Whirlpool di Napoli ha chiuso i battenti ha cessato le proprie attività. È stato chiuso, Ministro, dalla multinazionale che doveva garantirne la sussistenza, lasciando a casa centinaia di operai. I 355 impiegati dello stabilimento Whirlpool di Napoli avranno garantito lo stipendio fino al 31 dicembre, dopodiché il loro destino, il destino delle loro famiglie, il destino dei loro figli sarà incerto. sarà incerto. Nei giorni scorsi, insieme alle loro famiglie, ai sindacati e a tanti napoletani, hanno anche manifestato in una piazza storica di Napoli - Piazza Dante - per dare voce alle proprie difficoltà e per evidenziare le ricadute drammatiche che colpiranno non solo gli operai dell'azienda ma tutto il tessuto sociale del Meridione, del Sud. La chiusura dell'impianto Whirlpool di Napoli è il culmine della drammatica fase di impoverimento produttivo che investe ormai da anni il nostro Paese e che rischia di aggravare il quadro sociale ed economico del Mezzogiorno, del nostro Sud. L'intensa interlocuzione tra il Ministero e la multinazionale, purtroppo, non ha dato gli esiti dovuti e vorremmo sapere da lei, signor Ministro, se non ritenga doveroso adottare il prima possibile misure idonee atte a garantire l'adeguato supporto economico ai lavoratori dell'impianto della Whirlpool di Napoli, nonché se non ritenga opportuno istituire un tavolo di confronto presso il Ministero del lavoro al fine di poter trovare una soluzione che possa rilanciare lo stabilimento. Credo, signor Ministro, Credo, signor Ministro, che il Governo abbia il dovere di mettere in campo tutti gli sforzi necessari e possibili affinché si possa scongiurare un tale scenario, soprattutto in un momento drammatico come quello in cui stiamo vivendo. PRESIDENTE.

Ci sono poi gli investimenti in ricerca e sviluppo che sono misti tra fondo perduto e prestiti e che generalmente vengono concessi per finanziare nuovi prodotti e processi, quindi esattamente per questa finalità. benefici fiscali sotto forma di credito di imposta che possono essere applicabili agli investimenti in sito. C'è il nuovo fondo del MISE sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, quale possiamo utilizzare 10 milioni di euro tra *equity* e fondo perduto nonché i prestiti Sace che avrebbero potuto accompagnare questo percorso. Si tratta quindi di un pacchetto oggettivamente senza precedenti che è stato messo a disposizione di Whirlpool per restare. Quello che dico oggi è che, posto che gli stipendi sono garantiti fino al 31 dicembre, noi non dobbiamo trovare supporto economico agli operai che restano senza lavoro: dobbiamo trovare - e lo stiamo facendo - un imprenditore serio che voglia investire in quella fabbrica, e metteremo a sua disposizione tutti questi strumenti. Credo che la strada ci sia e le interlocuzioni che abbiamo in questo momento sono fondate e serie. Abbiamo fatto il possibile per fare stare Whirlpool a Napoli; oggi dobbiamo fare il possibile - e sono certo che ci riusciremo - per garantire che quelle persone non perdano il lavoro, ma che rimangano operative in quello stabilimento, anche se con un altro gruppo o con un altro prodotto.

mantiene fede agli impegni, quindi rimango speranzoso. Mi permetta però di dire che sarò soddisfatto e contento soltanto quando io e soprattutto gli operai della Whirlpool e i napoletani vedremo riaprire i battenti dell'azienda. I napoletani non hanno bisogno di sussidi, hanno bisogno di lavoro. Voglio ricordare ai miei colleghi che l'azienda Whirlpool, una settimana prima di essere chiusa, ha sfornato ancora prodotti tecnologici che fanno invidia al mondo. Ministro, la prego, non lasciamo gli operai della Whirlpool, i loro figli, le loro famiglie, nelle mani della manovalanza della criminalità. Lo Stato c'è, lo Stato siamo noi, lo Stato non deve essere disattento, perché quando lo Stato è assente, quando è distratto, ecco che l'anti-Stato sguazza.

che produce lavatrici. Ebbene, abbiamo capito che, dal 1° novembre, i lavoratori della Whirlpool (355) non producono più e hanno lo stipendio fino al 31 dicembre.

a quanto ha detto poc'anzi ricordando a tutti l'importanza del lavoro a Napoli: una città che rischia di esplodere delle tensioni sociali di questa seconda ondata di Covid che sta mettendo a dura prova la tenuta sociale e la tenuta democratica, perché nelle manifestazioni - legittime - delle categorie colpite dai DPCM soffiano i venti delle eversioni delle forze criminali. Questa classe operaia è pertanto un baluardo di difesa per la democrazia nella nostra città, nella nostra realtà. Attenzione, però, perché i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori

la stessa Whirlpool aveva investito e ci sono i *competitor* Candy ed Electrolux. Vado allora alla sostanza, Ministro. Lei ha detto che state lavorando a un progetto alternativo nella ricerca di un imprenditore di un imprenditore serio, ma siamo sicuri che non sia possibile riaprire una trattativa con la Whirlpool prima di procedere a questa ipotesi? Il 31 dicembre si sta avvicinando e quindi è incomprensibile il disimpegno. Sappiamo anche - me lo disse l'altra volta non abbiamo gli strumenti legislativi per poter far desistere da questa logica del "prendi i soldi e scappa". Proprio oggi depositeremo qui al Senato un disegno legge

senatore Ruotolo, che ringrazio per aver sollevato nuovamente il tema che è centrale, anche perché garantire il lavoro in una zona così difficile del Paese significa garantire che quelle persone siano lontane dalla criminalità e che non entrino in circoli viziosi molto pericolosi. Al di là del numero di persone coinvolte, il tema è di grande sensibilità e per questo ha attratto così fortemente l'attenzione del Governo e delle Assemblee parlamentari. Per una volta, mi permetto io di sollecitare il Parlamento a una discussione seria su una riforma che porti a dare strumenti al nostro Paese di protezione rispetto alle grandi aziende multinazionali che decidono di delocalizzare o di spostare le produzioni altrove. *(Applausi)*. È chiaro che il tema non può essere oggetto

o mille persone dipendenti e lo sforzo che viene chiesto all'imprenditore è di provare per sei mesi a trovare un'alternativa. Se non la trova, però, dopo i sei mesi di impegno non succede nulla. In realtà la penalizzazione del 2 per cento del fatturato avviene soltanto se si rifiuta di tentare di trovare una soluzione alternativa alla delocalizzazione. Credo che sia anche quella una norma molto debole e che vada invece fatto nel nostro Paese un ragionamento un po' più profondo. Credo che il tempo che abbiamo dedicato al tentativo di dare strumenti di convinzione e anche materiali a Whirlpool per restare ormai sia finito. Oggi dobbiamo essere certi di trovare una soluzione alternativa e io ci sto mettendo tutta la forza che ho per trovarla e vi posso assicurare che quel personale non starà un giorno senza uno stipendio.

apprezzo molto la sua risposta. Le chiedo ancora però, oggi che siamo al 12 novembre, di riprovare ad incontrare la Whirlpool con le organizzazioni sindacali per verificare la possibilità e le condizioni perché resti a Napoli. Quanto al progetto alternativo, è chiaro che a Napoli non serve assistenza ma serve questo. Dopodiché, è tempo che il Governo italiano apra questo *dossier* in sede europea, perché sappiamo poi che gran parte di questi dislocamenti di queste multinazionali finiscono nell'Est europeo; quindi c'è un tema di fiscalità, c'è un tema di salario

Signor Presidente, come il Ministro sa, la normativa sulle camere di commercio è stata oggetto di riforma a partire dal decreto legislativo n. 219 del 2016, che ha introdotto una serie di novità con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio fino alla loro *governance* complessiva. In particolare, l'articolo 3 dello stesso decreto ha previsto la riduzione mediante accorpamento del numero delle stesse camere di commercio, attraverso un decreto ministeriale che doveva essere attuato. Il decreto ministeriale doveva prevedere, in effetti, che le camere di commercio da 105 arrivassero a 60. Da allora un *iter* che si è successivamente prorogato ha portato purtroppo anche a numerosi ricorsi, a causa delle pesanti ricadute negative sulle imprese

tutte le conseguenze che possono ricadere sulle stesse industrie che, attraverso la camera di commercio, ricevono sostegno. Pertanto come parlamentari, credo, di tutte le parti politiche abbiamo presentato una serie di emendamenti

finalizzato a verificare, sulla base di criteri oggettivi, come promuovere un assetto più efficace. Ricordo infatti che lo scenario purtroppo è cambiato, c'è il Covid-19, quindi abbiamo ancora maggiore bisogno di sostegno per le nostre aziende. Pertanto, signor Ministro, siamo qui per chiederle quali atti lei abbia già prodotto per attivare questo tavolo e come stia procedendo l'*iter* per poter arrivare a un miglioramento delle nostre camere di commercio.

il nostro obiettivo è quello di avere camere di commercio efficaci ed efficienti, che diano servizi alle imprese. Certamente, restare appesi per quattro anni a una riforma non completata non è il modo migliore per raggiungerlo ed è per questo che in ogni occasione ho ribadito l'esigenza di portarla a termine, a prescindere dal tipo di riforma.

Percependo alcune criticità anche a livello territoriale, abbiamo inteso, nel decreto semplificazioni, con l'articolo 61, dare pari dignità alle sedi delle camere di commercio. Anche questo, infatti, non è un aspetto indifferente. Ritengo, quindi, che lo spirito del Parlamento e certamente quello Governo sia proprio quello di dare la possibilità alle camere di commercio di rappresentare

di tutti gli aspetti della riforma, ma soprattutto di come dare servizi migliori alle imprese, il tavolo sollecitato da un ordine del giorno proposto dalle Assemblee parlamentari è stato convocato per la giornata di lunedì 16 novembre

Signor Presidente, ringrazio il Ministro. Il Partito Democratico, come lei ben sa, come lei ben sa, considera fondamentale il ruolo delle camere di commercio per la funzione di prossimità e di aiuto che stanno dando alle imprese nei territori d'Italia, in questi mesi così difficili di crisi sociale ed economica causata, come sappiamo,

una soddisfazione per la sua iniziativa, che rende merito e dà continuità all'ordine del giorno che abbiamo approvato. Va quindi molto bene che il tavolo si apra; siamo convinti che non debba solo completare rapidamente una riforma con uno stile burocratico, ma che debba farlo con la logica sostanziale di completare una riforma soprattutto andando a vedere quali sono le eccezioni da correggere e quali accorpamenti vanno visti alla luce del seguente principio: noi vogliamo che sia valorizzato il patrimonio di storia, di tradizione e di buon governo di enti fondamentali dei nostri territori come le camere di commercio.

Gli effetti economici negativi hanno penalizzato soprattutto il comparto delle piccole, medie e grandi imprese, principalmente nel settore del turismo, dei trasporti, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato. A nostro parere, però, le scelte di questo Governo, che noi consideriamo dirigiste e stataliste, sono state orientate prevalentemente verso la nazionalizzazione delle società in crisi e la selezione di investitori sulla base del gradimento di Cassa depositi e prestiti, oltre a determinare una riduzione degli spazi di concorrenza

potrebbero essere più utilmente utilizzate se indirizzate a sostegno degli investimenti innovativi da parte di aziende piccole, medie e grandi e alla risoluzione di molte delle crisi aziendali che questa crisi pandemica e quindi economica ha generato riguardo alle piccole e medie imprese. Abbiamo bisogno di recuperare la fiducia dei nostri imprenditori e per farlo dobbiamo credere in loro, dobbiamo capire che evidentemente l'asse portante della nostra economia è proprio questa rete di piccoli, medi e grandi imprenditori che hanno basato le loro fortune sul loro coraggio, sulla loro voglia di investire,

sviluppo economico, quali stime abbia il MISE delle nuove crisi aziendali derivanti della situazione emergenziale e se, considerati i numerosi tavoli di crisi ancora aperti, stante la riacutizzazione dell'emergenza sanitaria e con essa il progressivo peggioramento della situazione economica del Paese, il Ministro non ritenga

quindi bisogno di qualche ora a disposizione per illustrare tutte le attività che stiamo svolgendo; in tre minuti cercherò di condensare alcuni elementi e spunti per rispondere alle giuste osservazioni e anche alle molte domande rivolte dagli interroganti, che ringrazio. Ricordo che abbiamo cercato di affrontare la crisi anche materialmente economica immediata rispetto alle chiusure, sia della prima fase che della seconda. Ad esempio, rispetto ai contributi a fondo perduto, che molto spesso sono denigrati, ricordo che abbiamo già erogato oltre un miliardo soltanto dell'ultima *tranche* del decreto-legge n. del decreto-legge n. 137, del 28 ottobre di quest'anno, quindi a distanza di dodici giorni abbiamo erogato oltre un miliardo di nuovi contributi a fondo perduto. Il decreto originale, che ha

Abbiamo previsto altri 2,2 miliardi con il cosiddetto decreto ristori e quasi un miliardo con il decreto ristori-*bis*. Ciò soltanto per affrontare un'emergenza di liquidità immediata soprattutto della piccola impresa.

per renderlo di durata certa e dare garanzia all'impresa di poter investire con serenità. Per quanto riguarda i tavoli di crisi, non esiste una norma, come ho detto più volte nelle Aule parlamentari, che stabilisca quando una crisi aziendale diventa un tavolo di crisi. Molto spesso c'è la

e al momento sono 795; certamente un numero molto pesante, ma siamo riusciti, soprattutto grazie all'azione del sottosegretario Todde, ad arrivare da 6.200 a 795 e riteniamo che ci siano ancora margini. Penso alla Ferriera di Servola, l'impianto siderurgico della mia città, dove si passa da 140 a 338 addetti nell'area a freddo. Penso ancora al percorso fatto per Embraco, una questione finalmente risolta con l'intervento di Acc. Sono state chiuse quindi molte vertenze

come spendere, ma a come investire le risorse che arrivano dal *recovery fund*. Al riguardo il lavoro che stiamo svolgendo al Ministero dello sviluppo economico è un lavoro intenso, che cerca di entrare in profondità rispetto alle fragilità dei nostri sistemi produttivi. intervenire in replica il senatore Pagano,

il Ministero non ha reso applicabili i decreti attuativi. Mancano decreti attuativi e quindi molti di quei danari che dovrebbero essere distribuiti alle imprese di cui parlavo prima, purtroppo non sono arrivati. È questo il dato. Il fatto che poi lei abbia fatto cenno ad alcune soluzioni di crisi aziendali, ci fa ovviamente piacere, spetta al suo Ministero occuparsene, ma è chiaro che quello che a me interessava di più era un vero e proprio piano rivolto al futuro che possa dare l'idea che l'Italia sta guardando verso il futuro con una visione. Lei ha fatto cenno al *recovery fund*, benissimo; come lei sa, noi abbiamo un'impostazione di tipo collaborativo. Forza Italia ha questo tipo di approccio. Noi le offriamo oggi,

recupero; troviamo il modo affinché il suo Ministero, che con lei soltanto non è in grado di farlo, possa dare delle risposte complessive. Chissà che magari anche col nostro contributo non sia possibile farlo.

depauperamento del sito produttivo, con lo spostamento di ordini verso altri siti aziendali, il tutto nel completo disinteresse dell'azienda, che non ha mai trattato la questione in maniera seria.

La giustificazione che è stata data è risibile: la denuncia dell'ultima trimestrale in rosso, in tempi di pandemia mondiale, è semplicemente un *escamotage.*

Questo è uno dei rari casi in cui un'azienda straniera arriva in Italia con una spregiudicatezza imprenditoriale mai vista prima, che sicuramente va fermata in quanto è anche a sfregio della della Costituzione italiana e dei suoi articoli 41 e 42, che ovviamente non è il caso di ripetere in quest'Assemblea. Ci chiediamo se non sia il caso di informare il nostro commissario europeo per l'economia Gentiloni per far conoscere a tutti quello che succede nella nostra

in suo potere e nelle sue competenze per evitare l'annunciata messa in liquidazione, attraverso un passaggio che è stato già fatto molto spesso sui suoi tavoli, ossia lo scorporo del ramo d'azienda ternano, così garantendo la prosecuzione dell'attività di questo sito e il

proprio nell'interlocuzione con chi nel territorio ci vive, così ottenendo maggior successo rispetto agli imprenditori, anche locali. Ritengo che sia assolutamente deprecabile l'atteggiamento dell'azienda. Noi chiediamo esattamente le cose richieste dai senatori interroganti, cioè che si possa arrivare allo scorporo di quella parte di attività, al fine di trovare una soluzione alternativa per continuare la produzione a Terni, visto che la situazione di Battipaglia è in realtà molto diversa. Siamo rimasti dunque oggettivamente basiti dal comportamento dell'azienda, che non ha accolto in minima parte la proposta e ha semplicemente comunicato unilateralmente la messa in liquidazione. Il sottosegretario Todde, che segue il tavolo, mi tiene costantemente informato. Credo che, in qualsiasi momento ci sarà un mio intervento diretto,

ci troviamo ad affrontare tematiche complicate e difficili, soprattutto in questo momento, non solo per la Treofan, come lei ha già detto, ma per tante altre aziende e noi parlamentari dobbiamo essere lì

Come possiamo essere i portavoce dei nostri territori, se dobbiamo ricorrere alle interrogazioni e non possiamo conferire, dialogare e discutere durante queste riunioni, che sono l'unico momento di confronto?

- Premesso che: la pandemia del COVID-19 ha colpito il mondo come un meteorite, spingendo l'economia globale nella peggiore recessione dai tempi della seconda guerra mondiale, danneggiando consumi, investimenti e paralizzando un numero crescente e inimmaginabile di attività, settori e mercati; invece, che ci si trova davanti a una grande sfida, che impone di realizzare politiche adeguate a sostenere e rilanciare l'economia e il livello di vita delle collettività; considerato che: in questo contesto il Governo, nell'avviato percorso del *green new deal*, si è impegnato a stimolare la ripresa consentendo all'economia di continuare a creare valore, puntando su un pilastro portante come il settore dell'edilizia; per dare nuovo impulso all'edilizia privata, grazie al Movimento 5 Stelle, il Governo ha recentemente introdotto la ben nota misura del "*superbonus*" uno strumento di rilancio e di sviluppo sostenibile che consente di effettuare lavori di miglioramento antisismico e di efficientamento energetico, ottenendo una detrazione fiscale superiore alla somma spesa per i lavori; per rendere ancora più efficiente ed efficace il "*superbonus*", ai fini del rilancio dell'economia, il contribuente può optare per lo sconto totale in fattura ovvero, in caso di impossibilità del committente di usufruire interamente della detrazione fiscale, la misura prevede la cedibilità di un credito di imposta di pari importo a qualsiasi altro soggetto, intermediari finanziari inclusi, e ancora la sua messa in circolazione senza limitazione numerica dei passaggi; da un'analisi compiuta da Unioncamere-Infocamere a livello nazionale è emerso che tra luglio e settembre 2020, grazie a questa misura, sono nate 4.971 nuove imprese edili, per tre quarti costituite da piccole realtà individuali, specialisti nelle attività di impiantistica, finitura degli edifici, posatori di infissi, espressione di una piccola e media impresa che è la spina dorsale del sistema produttivo italiano; Unioncamere ha ribadito che il "*superbonus*" al 110 per cento sta giocando un ruolo cruciale sulla vitalità del settore delle costruzioni che, sempre tra luglio e settembre, ha avuto un incremento dello 0,6 per cento su base trimestrale, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2019, da un sondaggio commissionato da "Facile.it", più di 21 milioni di italiani, l'equivalente di oltre 9 milioni di famiglie, hanno intenzione di utilizzare il *superbonus*, numero idealmente suscettibile di un ulteriore aumento in considerazione dei 14 milioni di famiglie che vivono nel milione di palazzi condominiali stimati sul nostro territorio nazionale;

specie nel caso di interventi di miglioramento antisismico, le cui procedure autorizzative potrebbero fortemente inficiare la sua reale attuazione, si chiede di sapere: se siano state avviate iniziative per estendere la durata del provvedimento oltre l'attuale scadenza di dicembre 2021, al fine di stabilizzare e rendere duraturi i benefici della misura sui territori; misura sui territori; se si intenda ampliare la possibilità di misura anche ad altri casi di protezione dell'ambiente, quali la riduzione di classi di rischio idrogeologico e misure volte al risparmio, riuso e riciclo della preziosissima risorsa idrica; se sia in in programma l'allargamento della platea dei beneficiari anche alle strutture ricettive e alberghiere, fra le più colpite dalla pandemia, per permettete al settore del turismo una ripresa vivace e pronta, attraverso una riconversione *green* dell'edilizia .

Credo che aver introdotto il superbonus riesca a farci raggiungere tre obiettivi distinti, tutti e tre importanti per il nostro Paese: dare fiato a un comparto, quello dell'edilizia, che è in crisi dal 2008, portare a un forte efficientamento energetico e a una maggiore protezione sismica del nostro tessuto immobiliare ormai datato e far sì che, grazie alla cedibilità del credito, anche le famiglie meno abbienti possano vivere in un appartamento e in un edificio più confortevole e più sicuri. Credo che questi siano obiettivi molto importanti, che vengono raggiunti da questo strumento che il MoVimento 5 Stelle ha tanto voluto e che ringrazio per aver spinto anche nella scorsa legislatura. È evidente che lo spettro temporale che abbiamo davanti rispetto a questa misura è troppo stretto e troppo stringente; stiamo lavorando proprio per ampliarlo. Non voglio dare dati o numeri, ma è certamente intenzione del Governo e immagino di tutto il Parlamento e di tutte le forze politiche sostenere la necessità di un prolungamento della misura. Rispetto alle proposte di ampliamento della stessa che gli interroganti hanno avanzato, ritengo che certamente possano essere introdotti nuovi interventi che siano anche trainanti. Penso che la risorsa idrica sia da tutelare, ma ritengo più difficile il ragionamento sul dissesto idrogeologico, che riguarda molto spesso ampie fasce di territorio e non un singolo immobile.

quindi bisognerà mirarlo rispetto ad altre forme incentivanti nei confronti di settori come il turismo, perché vi sono già strumenti sul campo che possono essere utilizzati dalle aziende del settore. Il dibattito parlamentare sulla legge di bilancio porterà magari a introdurre elementi rispetto al testo originale. Credo si debba ragionare anche su una razionalizzazione di tutto il sistema dei *bonus*, che si sono stratificati dal 1987 in poi. Il Governo su questo sta lavorando in modo serio e con efficacia. Signor Ministro, siamo naturalmente soddisfatti dei ragguagli che ci ha fornito. Il MoVimento 5 Stelle, sin dal principio, ha riconosciuto in questa misura *shock* una grande forza e ringraziamo sia lei che il ministro Fraccaro per aver lavorato molto su questo tema. una novità che, ancora prima che fosse attivo questo decreto, già quasi 5000 aziende, da luglio a settembre, si fossero attivate nel mercato dell'edilizia. È un dato molto importante. In un momento di crisi come questo, un provvedimento può essere un volano importante e impareggiabile, sia per i posti di lavoro sia, soprattutto, per il PIL che può generare a livello nazionale. È, però, fondamentale, sia sulla base pluriennale che sull'allargare i benefici, un'azione che avete portato quale avete aggiustato il tiro. È molto importante che si prosegua. Ha citato anche il *recovery plan*, che è uno degli spazi all'interno dei quali si può lavorare per rendere questa misura strutturale. Da riminese, sono molto sensibile all'accesso alle misure per le strutture alberghiere e ricettive. Sappiamo che le risorse sono poche in questo momento, ma dobbiamo trovare un varco importante perché il turismo abbia una possibilità di poter ripartire con questa manovra a fronte di una difficoltà molto grande che affronterà nel periodo 2020-2021. Dovremmo

Colleghi, ricorre oggi il triste anniversario dell'attentato di Nassiriya. Era il 12 novembre 2003 quando un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti all'ingresso della base italiana, nell'ambito della missione Antica Babilonia, provocando la morte di diverse persone, tra carabinieri, militari e civili. Quello che avvenne in quella tragica mattina è ancora ben vivo nella memoria di tutti noi. Ricordiamo ancora come tutto il popolo italiano fu scosso da un'ondata di addolorata partecipazione, con centinaia di persone che sfilarono dinanzi alle bare dei caduti esposti nel sacrario delle bandiere del Vittoriano. Oggi, come allora, il Senato si stringe attorno ai caduti per i valori di democrazia e solidarietà che contraddistinguono la nostra comunità nazionale. Osserviamo un minuto di silenzio.

desidero portare all'attenzione dell'Aula e del Governo l'ennesima mancata prevenzione, che ha riguardato catastrofi e disastri (ieri ci sono stati arresti

che hanno funestato l'Italia negli ultimi decenni, con migliaia di morti, seppur non paragonabili a quelli del Covid-19, questa disgrazia planetaria che ha contagiato oltre un milione di italiani, con quasi 43.000 morti. Mi riferisco, in particolare, al piano pandemico nazionale, che doveva essere aggiornato, ma che non è stato aggiornato. Con altri senatori del MoVimento 5 Stelle abbiamo depositato l'interrogazione

hanno aperto e poi richiuso, perché del tutto inutile. Lo aprimmo e lo buttammo nel cestino dopo due minuti. Il Paese ha pagato un prezzo molto alto per questo. Quel piano non entra nei dettagli. Invece, quello che fai in questi momenti dipende proprio da queste cose. ti prepari in base agli scenari: le terapie intensive, le mascherine. Quello del Ministro della salute era un piano che a livello operativo valeva zero». Signor Presidente, Presidente, il generale Pierpaolo Lunelli, ex comandante della scuola per la difesa nucleare, batteriologica e chimica, che ha contribuito a scrivere i protocolli militari contro la pandemia per alcuni Paesi e che ha stilato un rapporto indipendente di 60 pagine depositato in procura a Bergamo, ha dichiarato che se avessimo avuto il piano pandemico aggiornato,

che si chiama Ranieri Guerra, ma non è stato fatto. Le stragi non possono restare impunite. Anche se questa pandemia

il Governo deve rispondere.

straordinaria vicenda è lo stesso al quale si vogliono affidare addirittura i vaccini Covid. Io sono veramente molto preoccupato per questo, ma poi tanto non si risponde alle interrogazioni. Il 18 agosto ho presentato l'interrogazione

presso il quale si recava anche un certo Gesù di Nazareth, che chiedeva che fosse accettata la sola denominazione e connotazione culturale araba, cioè Haram al-Sharif.

Governo non vuole rispondere. Forse perché non può, forse perché vuole continuare, devo dedurne, a finanziare gruppi terroristici. È una cosa vergognosa e io denuncio la violazione del Regolamento del Senato.